dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori, su una strategia mondiale per il settore alimentare. Ha facoltà di parlare la senatrice Bertuzzi per illustrare la mozione n. 417.

è collegata ad un evento contingente, ma anche ad un vuoto politico non sopportabile in questo contesto. La contingenza corrisponde al vertice dei Ministri dell'agricoltura del G20, riuniti a Parigi, che tra oggi e domani dovranno esprimersi sui temi contenuti nel testo della mozione, e il vuoto politico corrisponde di fatto alla mancanza di una posizione ufficiale del nostro Paese, che il ministro Romano dovrà esprimere e che, per assenza di dibattito e confronto nel Paese, a tutt'oggi non ci è dato conoscere. Vi è una grande attesa su quelle che saranno le determinazioni del vertice: da un lato, vi è il diritto delle persone al cibo necessario alla sopravvivenza e il dovere dei Governi di assicurarlo; dall'altro, vi sono i produttori impoveriti da cause da loro non dipendenti che rischiano di allontanarli dalla loro missione principale, ossia la produzione del cibo. Quindi, da un lato, una domanda di cibo che aumenta e continuerà ad aumentare, visto il *trend* di crescita della popolazione mondiale e il cambiamento delle abitudini alimentari anche dei cittadini più abbienti dei Paesi emergenti; dall'altro lato, un'offerta di alimenti la cui produzione è minacciata dai cambiamenti climatici, dalle dinamiche di formazione dei prezzi delle derrate alimentari (che dipendono più dai mercati finanziari e dall'uso speculativo dei loro strumenti derivati che dal mercato reale dei prodotti), dalla mancata trasparenza negli *stock* di materie prime dei Paesi sviluppati, da un progressivo accaparramento delle terre dei Paesi poveri, dalla progressiva erosione dei redditi degli agricoltori. Nel corso di questa legislatura, la rincorsa delle emergenze economiche e sociali del settore agricolo ha esaurito i modi e i tempi della discussione, nascondendo di fatto la mancanza di una strategia capace di definire e guidare la *mission* dell'agricoltura del nostro Paese in modo chiaro e di concorrere, oggi, con forza alla risoluzione del vertice, chiamato ad un'assunzione di responsabilità collettiva dell'obiettivo lanciato nel 2000 dall'Assemblea delle Nazioni Unite, ossia di dimezzare entro il 2015 il numero delle persone che soffrono per la mancanza di cibo e che a tutt'oggi sembra molto lontano dall'essere raggiunto. Altrettanto elevate sono le preoccupazioni legate al pericolo che, nelle paure di una produzione alimentare presunta insufficiente, possano prevalere gli egoismi nazionali, preludio di un neoprotezionismo miope di fronte alla forza delle dinamiche globali. È evidente che le politiche poste in essere nei Paesi in via di sviluppo non sono state efficaci, ma è vero pure che le medesime dinamiche che hanno impoverito gli agricoltori hanno agito anche nell'aumentare il numero delle persone cadute in povertà. Si pone quindi per il nostro Paese, come nel resto del mondo, una rinnovata questione legata alla disponibilità di cibo, che trascende la questione settoriale e richiama ad un riavvicinamento dei cittadini e delle comunità ai produttori, in un protagonismo che riconosca questi ultimi come i garantì dell'offerta di cibo e della sicurezza alimentare. Come i padri fondatori della Comunità europea nella ricostruzione dei Paesi dopo la grande guerra compresero che la sussistenza alimentare delle popolazioni era il presupposto per far ripartire lo sviluppo economico e, prima ancora, sociale, e posero l'agricoltura come collante del patto sovranazionale, così oggi sfamare le popolazioni in un contesto mondiale richiama la costruzione di un patto internazionale, i cui confini abbracciano la dimensione globale degli scambi. Ci sono oggi le condizioni perché i Governi definiscano, attorno agli obiettivi delle Nazioni Unite, una comunità internazionale che superi le divisioni tra Paesi donatori e Paesi poveri e che costruisca una politica globale del cibo. La cultura del cibo locale, che si sta diffondendo nel nostro, come in altri Paesi, connessa ad una incalzante richiesta dei cittadini di sostenibilità ambientale, vivibilità dei territori, sicurezza degli alimenti, porta in sé un forte potenziale di innovazione sociale, che potrà esprimersi al meglio se si avrà la lungimiranza di interconnetterla con una dimensione globale del cibo, riempiendo di contenuti sociali i rapporti economici. L'accesso al cibo per tutti, la liberalizzazione dei mercati, il riconoscimento reciproco delle diversità agroalimentari, la domanda di partecipazione nei Paesi in via di sviluppo, l'innovazione tecnologica, la sostituzione dell'energia fossile con quella rinnovabile sono gli obiettivi in cui declinare la sfida lanciata dalle Nazioni Unite per superare i limiti e le inefficienze di una politica degli aiuti unilaterale. Il nostro Paese può e deve farsi promotore ancora una volta di una politica che riconosca al cibo una nuova centralità, contribuendo alla costituzione di una *partnership* globale sui temi dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e della nutrizione, che rilanci le istituzioni internazionali, promuova la conoscenza e l'innovazione come motori dello sviluppo, rafforzi il quadro giuridico internazionale sul reciproco riconoscimento dei sistemi di protezione della qualità dei prodotti, regolamenti i mercati finanziari per proteggere il cibo dalle mire speculative, fissi linee strategiche sugli investimenti nei terreni agricoli dei Paesi in via di sviluppo, sullo sviluppo rurale e sulla stabilizzazione dei prezzi sui mercati alimentari, coordini i sistemi di incentivazione delle fonti energetiche alternative. Ecco allora che anche il vuoto strategico nella politica nazionale trova una declinazione che ricolloca l'agricoltura al centro dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese. I confini delle strategie per il settore agricolo sono quindi molto più ampi e presuppongono coerenza con il contesto internazionale in un rinnovato rapporto tra produttori e consumatori-cittadini, ove la disponibilità del cibo e la sicurezza alimentare risultino questioni che non riguardano solo i produttori, ma l'insieme dei cittadini e delle comunità. È quindi importante che l'Italia si ponga alla testa della costruzione di una politica globale del cibo, sia in Europa che nelle relazioni internazionali, con il supporto magari trasversale di tutte le forze politiche presenti oggi in quest'Aula, così come hanno fatto le organizzazioni agricole italiane che hanno sottoscritto venerdì scorso, a Parigi la risoluzione finale di un *summit* che ha raccolto gli agricoltori provenienti da 75 Paesi in 120 organizzazioni. Per questo, auspichiamo il voto convinto favorevole di quest'Aula.

Signora Presidente, la fame nel mondo e in particolar modo nei Paesi sottosviluppati da sempre rappresenta uno dei problemi principali a cui le organizzazioni internazionali, quelle riconosciute a livello organizzativo e governativo, e il mondo cattolico, attraverso le organizzazioni dei missionari, hanno cercato di far fronte. La Dichiarazione La Dichiarazione del Millennio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre del 2000, impegna la comunità internazionale a sostenere la realizzazione, entro il 2015 e quindi a breve, di otto obiettivi prioritari attraverso un patto tra Paesi ricchi e Paesi poveri, finalizzato a costruire un mondo più prospero e più equo per tutti. Il primo degli obiettivi fissati è «sradicare la povertà estrema e la fame» e quindi dimezzare il numero delle persone il cui reddito è inferiore ad un solo dollaro al giorno. Dai dati in possesso alla FAO, nel 2010 il numero di persone sottonutrite è sceso a 925 milioni di persone, rispetto al miliardo e 23 milioni del 2009, e le stime per il 2011 indicano che tale numero diminuirà ancora a livello globale, in maniera diversificata nei vari Paesi in via di sviluppo. Il problema della fame nel mondo rimarrà concentrato nell'area dell'Asia, del Pacifico e soprattutto in quella africana. Nonostante sia prevista questa diminuzione (la prima negli ultimi 15 anni), il numero delle persone estremamente povere rimane a livelli inaccettabili e inammissibili. Pertanto, è ancora più urgente la necessità di individuare soluzioni alla carenza di prodotti agricoli e alimentari e alla distribuzione delle stesse risorse tra Paesi ricchi e Paesi poveri. La sopravvivenza delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo dipende quasi esclusivamente dall'agricoltura. Lo sviluppo rurale di regioni povere svolge un ruolo essenziale nel promuovere la produzione e la sicurezza alimentare, combattendo fame e malnutrizione, che sono diffusissime. In gran parte dei Paesi in via di sviluppo, l'agricoltura è ancora essenzialmente di piantagione, assorbe la maggior parte degli investimenti e produce solo per 1'esportazione.

Si può produrre molto anche dove di acqua ce n'è poca: basta vedere le esperienze sicuramente positive del popolo israeliano, che vive certamente in una terra ostile ma, nonostante questo, riesce comunque Non possiamo continuare con le monocolture, perché queste penalizzano ulteriormente lo scambio

I fattori che influenzano la capacità delle economie rurali di garantire la sussistenza alle loro popolazioni sono molti e riguardano fenomeni interni ed esterni al mondo dell'agricoltura, quali l'accesso alla terra e il controllo e la gestione delle risorse locali; i cambiamenti climatici, che incidono sulle rese agricole - è evidente - e comportano la volatilità del prezzo globale degli alimenti, causato

degli squilibri nel sistema globale di approvvigionamento alimentare; l'intensificazione dell'uso dei prodotti agricoli per la realizzazione di biocarburanti ha fortemente alterato il mercato agricolo:

in etanolo. Anche in Brasile, gran parte del terreno agricolo viene utilizzato per produrre energia, principalmente bioetanolo estratto dalla canna da zucchero,

in due anni. Credo che questo sia un motivo di profonda riflessione da parte di tutti. È evidente quindi come l'agricoltura e la produzione di cibo svolgano un ruolo primario nel processo di riduzione ed eliminazione della povertà estrema. Lo sviluppo rurale dei Paesi in via di sviluppo non può prescindere

In molti Paesi in via di sviluppo le donne - lo sappiamo - risultano vitali per la produzione alimentare. Su questo tema, sia la FAO sia noi sosteniamo la tesi che, diminuendo le disuguaglianze e le discriminazioni nei confronti delle donne, automaticamente aumenterà la forza

principali motivi che hanno recentemente fatto scoppiare parecchie guerre nel Nord Africa, con le conseguenze che tutti quanti conosciamo. All'attuale modello della produzione intensiva, la Divisione produzione vegetale e protezione delle piante della FAO oppone un nuovo modello mirato alla preservazione, ovvero a un insieme di tecniche dell'agricoltura di conservazione e precisione nella coltivazione. Le prime consistono in una serie di pratiche agronomiche in grado di limitare gli effetti negativi sulla composizione del suolo, mentre con un'irrigazione e un impiego di fertilizzanti più preciso (e più ecologico), si potrà produrre di più con meno acqua e raddoppiare l'ammontare di nutrienti assorbiti dalle piante. Completa la strategia un metodo per combattere i parassiti senza un eccessivo ricorso ai pesticidi (quindi si pensa all'agricoltura biologica). La FAO fa sapere che, oltre ad accrescere la produzione di cibo, queste tecniche contribuiscono a ridurre il fabbisogno di acqua del 30 per cento e i costi energetici fino al 60 per cento, permettendo in alcuni casi di incrementare di ben sei volte le rese agricole.

attrarre i meccanismi nazionali di selezione delle specie vegetali e fornire incentivi all'adozione di questo nuovo modello. Lo studio auspica infine un aumento generalizzato degli investimenti nell'agricoltura, soprattutto da parte dei Paesi sviluppati cui si chiede di aumentare la quota di aiuti ufficiali allo sviluppo

che, di fatto, hanno mantenuto il precedente sistema di sfruttamento della popolazione osteggiando l'iniziativa privata e consentendo a poche élite di godere dei profitti derivanti dall'economia. Signora Presidente, concludo dicendo che è necessario dare a questi Paesi, oltre che i soliti finanziamenti, che spesso e volentieri non sappiamo che fine fanno, gli strumenti per poter lavorare e poter costruire a casa loro. Credo che un motivo di riflessione sia un vecchio e saggio detto popolare che a noi della Lega Nord sta molto a cuore e che condividiamo, il quale dice che per aiutare le persone che hanno fame è giusto e corretto dare loro la vecchia barca - nel senso metaforico del termine - con alcune canne da pesca e insegnare loro a pescare, e a pescare bene, piuttosto che regalare loro qualche chilo di pesce.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, i Ministri dell'agricoltura del G20 si riuniscono oggi e domani a Parigi: sul tavolo hanno la crisi alimentare cui sta andando incontro il Pianeta e, appena fuori, in un grande e sviluppato Paese come la Francia, la siccità sui campi e l'esaurimento delle risorse ittiche nei suoi mari. Ringrazio la collega Bertuzzi e gli altri firmatari della prima mozione in discussione, che con la loro iniziativa consentono oggi questo dibattito nell'Aula del Senato, tardivo certamente rispetto al G20 ma necessario, si spera, per influire sulle politiche del Governo italiano, anche in sede internazionale. È quello che tentiamo di fare con la nostra mozione, che riporta i dati allarmanti della fame nel mondo e le stime, tragiche, di un pianeta sempre più sterile ma con una popolazione in crescita, 9 miliardi nel 2050. Da un decennio assistiamo al lento ma costante aumento della fame cronica (sono 925 milioni gli affamati nel mondo, il 98 per cento dei quali vive nei Paesi in via di sviluppo), e proprio a poco più di dieci anni fa risale la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, che impegna i 191 Stati membri a raggiungere, per l'anno 2015, otto obiettivi, il primo dei quali è sradicare la povertà estrema e la fame che invece in questi dieci anni è aumentata: nei Paesi in via di sviluppo, ma soprattutto in un grande Paese emergente come l'India, e nei cosiddetti Paesi sviluppati. Le responsabilità coinvolgono le politiche e i Governi, e le industrie del settore. Il Pianeta è in marcia verso il disastro alimentare, e noi vorremmo anche il nostro Paese impegnato a evitare una crisi che vede un essere umano su sette ridotto alla fame ogni giorno, pur vivendo in un mondo capace di nutrire tutti. Ricordo qui il paradosso con cui si apre lo *State of the World* 2011 del *World Watch Institute*, che si intitola proprio «Nutrire il Pianeta» ed è stato scritto da esperti mondiali del settore agricolo: «Viviamo in un mondo in cui si produce più cibo che mai, ma dove gli affamati non sono mai stati così numerosi». Basti pensare a un dato, impressionante, che il rapporto evidenzia: per cento del cibo prodotto annualmente in tutto il mondo viene sprecato prima di essere consumato. Insomma, il Pianeta è sempre più sterile e affamato, e lo è perché sempre più folle. Noi vorremmo che l'Italia, che del resto, come la Francia prima citata, è vittima della siccità e della desertificazione, ed è terra d'approdo per chi fugge dalla fame e dai Paesi in rivolta del Nord Africa, si attivasse in Europa e nell'ambito delle relazioni internazionali perché emerga, nei fatti oltre che negli impegni, la più ampia e condivisa determinazione al fine di evitare la crisi alimentare alle porte. Che cosa si può fare e subito? Intanto dare ascolto e sostegno alle soluzioni che, pur partendo da approcci diversi, propongono, per esempio, sia la FAO sia il *World Watch Institute* e che nella nostra mozione sono richiamate: oggi più che mai c'è bisogno di un'agricoltura che sappia produrre preservando, conservando la fertilità dei suoli e acqua e aria pulite; in più bisogna cambiare il modo in cui gli alimenti sono trasformati e commercializzati; si devono considerare, e riconsiderare, i tipi di imprese nel settore alimentare in cui si sta investendo. Per fare questo, impegniamo il Governo a promuovere il sostegno agli agricoltori, in particolare dei Paesi in via di sviluppo, perché possano apprendere e applicare nuove pratiche agricole e tecnologie già ampiamente sperimentate, quelle in particolare che consentono di preservare le risorse naturali. I Paesi sviluppati devono incrementare la quota di aiuti ufficiali all'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo, non per sostenere le multinazionali del settore o Governi corrotti che si alimentano della fame dei loro popoli, ma con incentivi all'adozione di quei modelli produttivi che esistono, e gli studi citati nella mozione ne danno ampia dimostrazione - che capitalizzano le risorse naturali senza depauperarle. Proprio dal G8 riunito all'Aquila nel 2009 è partita una grande iniziativa per la sicurezza alimentare che oggi segna il passo: deludente è stato a tal proposito il recente G8, da cui non sono scaturite misure concrete per garantire lo stanziamento dei fondi promessi due anni fa all'Aquila. L'Italia, con il suo aiuto pubblico allo sviluppo pari allo 0,15 per cento, a fronte di un obiettivo dello 0,51 per tenacemente insistere per il rispetto degli impegni presi all'Aquila soltanto dopo che avrà riconquistato - e questo è importante - una credibilità internazionale. E a tal fine, oltre che stanziare i fondi dovuti, il nostro Paese deve frenare quello smantellamento della cooperazione italiana allo sviluppo in atto da tre anni. Gli investimenti del settore privato, che sembrano l'unica strada perseguita dal nostro Governo per le aree di crisi del mondo, rischiano di contribuire soltanto al disastro, se non subordinati e comunque guidati dalla volontà di raggiungere il primo degli obiettivi del Millennio, cioè sradicare la povertà estrema e la fame entro il 2015. Infine, ma fondamentale, l'ascesa dei prezzi delle materie prime agricole e degli alimenti: le cause sono molteplici e complesse (basti pensare che una di queste è proprio il maggior benessere nei Paesi emergenti, un'altra è l'aumento del costo del petrolio, ma al contempo anche la produzione di biocarburanti è complice di questa ascesa), il fenomeno sembra inarrestabile, tanto che ONU e FAO ripetutamente lanciano allarmi. La volatilità dei prezzi delle materie prime agricole può avere effetti negativi estesi sul settore dell'agricoltura, sulla sicurezza alimentare e sull'economia in senso più ampio, sia nei Paesi sviluppati, sia in quelli in via di sviluppo. È chiaro a nostro avviso che l'Italia, soprattutto nella Comunità europea, deve collaborare e incentivare a intervenire contro la speculazione, contro l'assenza di trasparenza e di regolamentazione nei mercati, tenendo però presente che il solo autentico freno alla speculazione verrà dalla presa in carico del Pianeta, dalla capacità di ricostituire le sue risorse, di fermare il cambiamento climatico, di ridurre almeno la folle crescita di obesità e rifiuti da una parte, e di desolazione e sradicamento dall'altra.

Signora Presidente, anche il Popolo della Libertà intende contribuire a questo dibattito con particolari accenti che riguardano la politica comunitaria e l'individuazione, sin qui ben esposta, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi della Dichiarazione del Millennio. In particolare, riteniamo che il blocco dei negoziati del WTO (*World Trade Organization*) abbia determinato in questi ultimi anni l'aumento della sperequazione tra la quantità e la qualità di derrate disponibili per i Paesi sottosviluppati, quelli in via di sviluppo e i cosiddetti Paesi che fanno che fanno dell'agricoltura di qualità una delle principali risorse finanziarie. Una sorta di veto incrociato tra questi Paesi ha impedito la libera circolazione delle derrate, ma soprattutto l'accumulo di derrate. Ricorderete tutti come quattro o cinque anni fa anche in Europa, anche in Italia, vennero esaurite le scorte di grano. Invece la necessità della diversificazione nella collocazione delle *commodities* è di straordinaria importanza. Pensiamo a Paesi come l'India, per esempio, dove non si faceva ricorso al mercato internazionale ma l'approvvigionamento avveniva in maniera molto diversa, anche con produzioni locali. Quindi, questo grande cambiamento, che ha determinato grosse speculazioni nell'accumulo e nell'accaparramento di derrate, non ha fatto altro che peggiorare la sperequazione e accentuare la fame nel mondo. In particolare, la nostra mozione vuole sottolineare come le le trattative in corso sulla riforma della PAC possono sicuramente incidere positivamente per il raggiungimento di questi obiettivi che ci siamo prefissi. L'Italia è stata sempre in prima linea, quando si parla di qualità alimentare, e in questo G20 sicuramente ciò sarà ulteriormente sottolineato. La qualità alimentare è diventata di straordinaria importanza. Negli anni scorsi molto spesso ci siamo chiesti se il ricorso agli OGM potesse risolvere o meno il problema della fame nel mondo incrementando le produzioni. Si sta raggiungendo una sorta di equilibrio su questo tema, nel quale, oltre alla quantità, è di fondamentale importanza anche il raggiungimento della qualità nelle produzioni. L'Italia tiene molto alla qualità dei suoi prodotti, e quindi va perseguita con sempre maggiore intensità una politica non protezionistica - non è questo ciò che vogliamo - ma sicuramente di valorizzazione della qualità dei nostri prodotti.

ha determinato nell'ultimo decennio un'inversione di tendenza riguardo alla loro destinazione. L'Italia,

di far sì che non venga ridotto il *budget* per la politica agricola comunitaria, ma che venga mantenuto e anzi incrementato, perché ciò è di fondamentale importanza anche per gli obiettivi del del Millennio, che l'Italia vuole sicuramente perseguire. Stiamo quindi discutendo nei fori internazionali su questo tema, al quale affianchiamo quello della contraffazione.

incide sulla qualità della vita. Inoltre, siamo convinti che l'agricoltura di qualità determina anche la qualità dell'ambiente. L'agricoltore deve recuperare - e ciò deve essere assolutamente sancito e riconosciuto da tutti quel fondamentale ruolo di tutore dell'ambiente che gli è da sempre riconosciuto, ma che forse una politica ambientalista un po' radicale ha in qualche modo

si riprendano i negoziati del WTO, che in sede comunitaria vengano stanziate le giuste risorse per la riforma della PAC, che sia garantita la qualità dei prodotti e che l'Italia comunque rimanga in prima linea per raggiungere gli obiettivi del Millennio.

«Pane e democrazia!», hanno gridato da piazza Tahir al Cairo, nello Yemen, ad Algeri, ad Amman; «Pane e democrazia!», hanno gridato donne e uomini su Internet, rinforzando il legame tra democrazia e comunicazione, un legame inscindibile, che prima o poi libererà non solo questi Paesi, ma forse anche l'Iran e la Cina. Lo ripeto per il collega e la Cina; perché noi che ci occupiamo della pace ci ricordiamo di questi Paesi anche quando non accadono fatti specifici. Spero che anche lui lo ricorderà nel suo prossimo intervento. E certamente questo legame unirà le forze di chi crede nella libertà e nell'uguaglianza ma sa che esse, senza la fraternità, sono destinate solo a dividere. E, pur gridando in Internet o nei media ormai globalizzati, non hanno smesso di ripetere questo grido di pane e democrazia, a ricordarci che la libertà va di pari passo con la libertà dal bisogno. Quando questa viene a mancare, non c'è secolo tecnologico o nuovo millennio che tenga. il ritorno di uno *slogan* antico che azzera fondamentalismi e teorie ideologiche. Nei Paesi del Nord Africa e del Maghreb, nei Paesi arabi mediterranei, le piccoli o grandi rivoluzioni che abbiamo visto accadere, che stanno accadendo e che accadranno ancora portano questo segno comune: la insostenibilità di una condizione che mortifica il corpo ma anche lo spirito. Come due o tre secoli fa, i prezzi alimentari, le condizioni economiche di una fase di passaggio epocale dello sviluppo, le speculazioni e le rendite sono state il detonatore di rivolte che, seppure localizzate territorialmente, interrogano il mondo intero. Un miliardo di esseri umani che rischiano la fame e la morte dei loro figli per fame; il 98 per cento della denutrizione e della fame concentrato nei Paesi in via di sviluppo; la tragica carambola dell'aumento del prezzo del carburante che serve per coltivare biocarburanti, che mangiano terra che dovrebbe servire a poter far mangiare gli stessi esseri umani proprietari, o solo affittuari, di quella stessa terra; infine*,* lo sfruttamento e il furto di terra buona e coltivabile, sempre più diffuso. Penso non all'Africa, a cui tutti pensano sempre, ma al Sud America, che si sta riprendendo da poco, dove le grandi compagnie internazionali OGM che noi condanniamo e dove comprano terre che appartengono ad altri. Tutto ciò e molto altro ritroviamo nelle contraddizioni di uno sviluppismo superato dal secolo scorso, di un consumismo che è una variante impazzita dello stesso capitalismo, poiché usa i capitali non per produrre beni, ma solo per moltiplicare profitti e beni immateriali. È o non è questa la grande questione non rimuovibile di cui stiamo parlando? Questo sistema, questo stato di cose, colleghi, non è inamovibile né ineluttabile. Serve una riunificazione delle forze in campo internazionale, serve una nuova iniziativa della FAO, che proprio in questi giorni eleggerà il suo nuovo direttore generale, a Roma. Serve una nuova strategia di coordinamento mondiale che non accetti di occuparsi, lodevolmente, di diminuire la fame nel mondo con i *Millennium goals* (i cui impegni peraltro il nostro Paese, come molti altri, non rispetta) rispetta) salvo poi voltare il capo quando si tratta di parlare di proprietà delle terre, uso consapevole di esse, commercio equo ed equi salari, investimento nella ricerca e nell'innovazione, commercio e mercato regolati e*partnership* di sviluppo tra Paesi produttori e non. In Africa, per la quale si piange troppo spesso retoricamente, solo il 27 per cento delle superfici coltivabili è veramente utilizzato e, su un potenziale di irrigazione di 42 milioni di ettari, ne è utilizzato solamente un terzo: altro che soddisfacimento delle condizioni date! Vedete, in questo senso c'è da svolgere un ruolo importante anche per il nostro Paese. Certo, si tratta della PAC, PAC, ma anche di un cambio di filosofia, in un settore - quello agroalimentare - che non è più solo economico, ma incide su bisogni, desideri, stili di vita e salute.

Il cibo sfama, ma costruisce anche comunità, crea simboli e ritualità, stabilisce relazioni umane, economiche e sociali. «Pane e democrazia!», chiedono i popoli in rivolta, non solo l'uno o solo l'altra. Illudersi che basti offrirli divisi, e non porsi il problema durevole del sistema economico mondiale e nazionale che stiamo costruendo, o dovremmo costruire, sarebbe un errore che faremmo pagare alle future generazioni. Colleghi, non c'è abbastanza pane per chi chiede libertà, non c'è abbastanza democrazia per chi viene sfamato nell'ingiustizia e nell'asservimento, e chi pensa che abbiamo parlato solo di prezzi e derrate alimentari continui pure a dormire tranquillo, quel grido nato a piazza Tahir, «Pane e democrazia!», continuerà a non sentirlo mai per quanta economia, anche agricola, possa aver studiato. richiamare l'attenzione dell'Aula in particolare su due aspetti. Il crescente conflitto tra l'uso delle derrate agricole per fini alimentari e per la produzione di biocarburanti e il riflesso sul diritto dell'accesso al cibo dell'uso speculativo

anche nei Paesi sviluppati, cresce il numero delle persone denutrite, che sono quasi 19 milioni. È il paradosso: un sistema agricolo che produce cibo sufficiente per alimentare 12 miliardi di persone ma ne lascia un miliardo senza sufficiente alimentazione, mentre nel mondo oltre un miliardo di abitanti è alle prese con i problemi di eccessi di cattiva alimentazione (obesità, diabete, problemi circolatori). II problema non è la mancanza di cibo, ma la sua cattiva distribuzione, e il fatto che una parte della popolazione mondiale non ha risorse sufficienti per poterlo comprare. Il picco dei prezzi agricoli del 2007-2008, dovuto anche a fenomeni speculativi, è destinato a ripetersi: l'OCSE stima per il prossimo decennio un aumento tra il 20 e il 40 per cento dei prezzi di mais, prodotti oleosi e zucchero. cento delle superfici coltivate è destinato all'alimentazione animale, e la diffusione degli allevamenti animali è una delle cause maggiori dell'aumento delle emissioni di CO2. Prezzi più alti non significano automaticamente prezzi più remunerativi per i piccoli produttori agricoli. Cinque grandi multinazionali controllano più della metà del nostro cibo attraverso il controllo su semi, pesticidi, fertilizzanti; l'accaparramento delle terre e il dominio sul mercato di grandi società emargina la rete dei piccoli produttori; cresce il costo dei principali fattori di produzione e si erode per loro il margine di profitto. La quantità di prodotti agricoli destinati alla fabbricazione di biocarburanti è in costante crescita. L'OCSE e la FAO nel loro rapporto annuale calcolano che al 2020 il 13 per cento della produzione di cereali secondari, cento della produzione di oli vegetali ed il 30 per cento della produzione della canna da zucchero siano destinate alla produzione di biocarburanti. C'è un legame ormai diretto tra prezzo del petrolio e prezzo dei prodotti agricoli. Si stima che una crescita del 25 per cento del prezzo del petrolio comporti una crescita del 5 per cento del prezzo dei cereali secondari e del 3 per cento per il grano e le piante oleose. Occorre perciò rivedere profondamente le politiche di incentivazione fin qui adottate; occorre selezionare biomasse che presentino rapporti elevati del rapporto energetico, buone rese produttive senza eccessivi apporti di acqua e sostanze chimiche; occorre indirizzarsi verso l'utilizzo di biomasse che non abbiano un valore alimentare o che entrino in modo del tutto marginale nella catena alimentare, per evitare fenomeni di rarefazione delle derrate alimentari e speculazioni sui prezzi con gravi effetti per i livelli alimentari dell'umanità; occorre, infine, valorizzare la coltivazione di aree agricole marginali o abbandonate, favorendo lo sviluppo di forme produttive associate. Sarebbe indispensabile introdurre in modo obbligatorio dei sistemi di certificazione indipendente che accertino la reale sostenibilità dei carburanti prodotti, sotto il profilo energetico ed ambientale, riservando unicamente a questi ultimi eventuali incentivi II secondo aspetto riguarda l'accresciuta volatilità dei prezzi agricoli a brevissimo termine, non più influenzati solo dall'andamento della domanda e da quello dell'offerta o da fatti straordinari, ma da un accresciuto afflusso di capitali speculativi. Anche il cibo entra nel grande gioco delle scommesse della finanza speculativa a livello globale. Le conseguenze sono una minaccia alla vitalità delle aziende agricole (prezzi troppo bassi) e alla sicurezza alimentare, quando i prezzi aumentano. I guasti prodotti dagli eccessi speculativi senza regole sul sistema finanziario rischiano di replicarsi sul sistema del cibo. Ritorna pertanto anche in questo campo il punto centrale: non si può globalizzare la finanza ed il commercio senza una corrispondente globalizzazione delle istituzioni politiche.

gli obiettivi di sviluppo del Millennio impegnano la comunità internazionale al conseguimento di importanti traguardi, primo tra tutti la riduzione della povertà estrema e della fame, il che equivale a dimezzare il numero delle persone il cui reddito è inferiore ad un dollaro al giorno, la maggior parte delle quali vive nei Paesi in via di sviluppo. Noi non possiamo che condividere tale ambizioso traguardo: il mondo deve sconfiggere la povertà estrema - soprattutto neonatale - e le malattie e innalzare la qualità della vita di ogni essere umano che abita il Pianeta; nonostante recenti dati FAO siano incoraggianti (evidenziando una riduzione del numero delle persone sottonutrite), la quantità di «estremamente poveri» rimane a livelli molto alti e pertanto è ancora più urgente la necessità di individuare soluzioni alla costante carenza di materie prime alimentari e alle disuguaglianze generate dalla ineguale distribuzione delle stesse tra Paesi ricchi e Paesi poveri. L'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli e la speculazione sul rialzo delle quotazioni di molte materie prime agricole, dovuto al mutamento dei sistemi di alimentazione delle popolazioni dei Paesi ricchi, non fanno che peggiorare una situazione già drammatica ed evidenziare ulteriormente gli squilibri del sistema di approvvigionamento alimentare. I cambiamenti climatici e i disastri ambientali - penso allo tsunami che ha colpito il Giappone - innescano inoltre processi a catena in cui l'aumento del prezzo di un bene provoca quello di tutti gli altri, specialmente dei beni alimentari, aggravando ancora di più le problematiche legate alla povertà estrema. La silenziosa crisi alimentare, che colpisce un sesto dell'intera popolazione mondiale, costituisce inoltre un serio rischio per la pace e la sicurezza nel mondo e i fatti accaduti gli scorsi mesi in Nord Africa sono l'esempio più recente. È noto che l'agricoltura rappresenta il fattore essenziale di sopravvivenza per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e pertanto lo sviluppo rurale delle regioni povere svolge un ruolo essenziale nel promuovere la sicurezza alimentare e combattere la fame e la malnutrizione; sono necessari però interventi strutturali che introducano correttivi agli attuali sistemi agricoli dei Paesi in via di sviluppo, caratterizzati dalla presenza di agricoltura di piantagione che assorbe la maggior parte degli investimenti e produce solo per l'esportazione e dal carattere monocolturale della stessa che penalizza ulteriormente la ragione di scambio e innesca processi di disequilibrio territoriale con conseguente maggior aumento della desertificazione e delle carestie. Possiamo citare l'esempio del Senegal dove le piantagioni di arachidi per esportazione occupano il 40 per cento delle terre coltivate ed assorbono la maggior parte degli investimenti; per incrementare ulteriormente le produzioni, in associazione con il Mali e la Mauritania, il Paese ha intrapreso una serie di grandi opere idrauliche sul fiume Senegal che, una volta ultimate, dovranno recuperare all'agricoltura monocolturale di piantagione oltre 500.000 ettari di terreni semidesertici. La frontiera agricola verrebbe quindi spostata verso l'entroterra settentrionale, innescando quei processi di disequilibrio territoriale che sono stati la causa della desertificazione e delle carestie degli anni Per contro l'agricoltura di sussistenza, che produce miglio, manioca e riso per il fabbisogno della popolazione, non riceve adeguati sostegni finanziari ed il Paese è costretto ad importare i generi alimentari di prima necessità. Dunque, noi riteniamo che l'insicurezza alimentare vada combattuta con interventi che mettano al centro dello sviluppo le popolazioni locali, che le rendano partecipi dei processi di miglioramento della propria condizione in un'ottica di sviluppo sostenibile nel tempo. La fame di parte della popolazione del mondo è inaccettabile e non può essere considerata una sorta di normalità che impegna i Paesi sviluppati a predisporre programmi di aiuto e di assistenza, il più delle volte gestiti da governanti corrotti che ostacolano spesso qualsiasi tentativo verso assetti istituzionali democratici. L'unica vera normalità può, infatti, essere un mondo in cui l'accesso al cibo e ad alimenti salubri, sufficienti e nutrienti, sia per tutti. Gli impegni da portare avanti, a nostro avviso, per una politica globale che assicuri il diritto al cibo, riguardano sia la necessità di aumentare la quantità e la qualità della produzione agricola, eliminando i fattori strutturali che possono incidere sulla volatilità dei prezzi delle materie prime, sia interventi che promuovano lo sviluppo rurale dei Paesi in via di sviluppo mediante azioni strutturali finalizzate ad aumentare la produttività, in particolare dei piccoli agricoltori che si collocano al di fuori del sistema dell'agricoltura commerciale e che devono essere messi nelle condizioni di poter beneficiare delle dinamiche dei mercati e di migliorare l'accessibilità ai servizi finanziari rurali che favoriscano la libera iniziativa. Riteniamo, inoltre, indispensabile rivedere il sistema dei finanziamenti alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative, alcune delle quali hanno perso di vista lo scopo per cui sono state create e sono molto più attratte dalle possibilità di guadagno offerte dalla cooperazione piuttosto che da scopi umanitari. È altresì indispensabile promuovere criteri di finanziamento basati sul conseguimento di obiettivi misurabili e di progetti sostenibili al fine di potenziare l'efficacia e la resa degli aiuti.

ha a che fare in maniera stringente con la qualità della globalizzazione a livello mondiale. La globalizzazione La globalizzazione all'inizio del secolo, circa 10 anni fa, veniva letta sostanzialmente come l'estensione imperialistica

di centinaia di milioni di esseri umani, già esclusi dallo sviluppo, dentro lo sviluppo stesso. Questo, che di per sé è un fatto straordinariamente positivo, naturalmente comporta una serie di problemi nuovi, con i quali dobbiamo confrontarci,

quando c'era un Primo, un Secondo e un Terzo mondo, quando c'era un grande Terzo mondo affamato di fronte a un Primo e ad un Secondo mondo che si contrapponevano tra loro secondo la logica dei blocchi. Questo mondo non c'è più, e quello con il quale dobbiamo fare i conti è un mondo completamente diverso, un mondo paradossale nel quale, sulla base dei dati delle Nazioni Unite, tra il 1990 e oggi,

sono diminuite di cinquecento milioni di unità. Siamo passati da un miliardo e mezzo di esseri umani che vivevano con meno di un dollaro al giorno a quasi un miliardo attuale. l'equivalente di due Europe nel mondo vive con meno di un dollaro al giorno, e questo è uno scandalo, dal punto di vista morale e politico, inaccettabile

riferisco a quante persone vivono la fame rispetto a quelle che vivono la povertà. Non esiste più un nesso immediato, automatico, perché le persone che vivevano in condizioni di sottonutrizione erano 840 milioni nel 2000

responsabilità. Vi dico, solo per titoli, i tre obiettivi che dovremmo raggiungere. Il primo è combattere il protezionismo nel mercato dell'agricoltura. Su questo, l'Europa ha molto da farsi perdonare. L'Europa, che giustamente sostiene le politiche umanitarie sul fronte degli aiuti, è all'avanguardia nel mondo delle politiche di cooperazione allo sviluppo, ma ciò che dà con una mano lo sottrae in maniera ancora più forte con l'altra, riducendo drasticamente l'accesso

e naturalmente la disincentivazione dell'uso delle aree agricole per la produzione di carburanti. Credo che su questo il Governo italiano debba fare di più di quanto sta facendo. Credo sia giusto che il Parlamento, e il Senato in prima linea, lo spinga e lo solleciti in questa direzione.

c'è da dire che, indubbiamente, il cibo rappresenta un elemento centrale della vita degli individui per i suoi molteplici significati, per la sua disponibilità e per il fatto che costituisce un diritto fondamentale per tutti i cittadini del mondo. Tuttavia, ad oggi, assistiamo al fatto che molti Paesi in via di sviluppo non sono ancora riusciti a dotarsi di politiche efficaci e di piani che possano aumentare gli investimenti e promuovere il diritto all'alimentazione per i propri cittadini. I cambiamenti climatici, l'innalzamento dei prezzi degli alimenti ed il mutamento dei modelli di consumo nelle fasce più ricche della popolazione dei Paesi emergenti determinano problemi che potrebbero influire negativamente nei processi di crescita di quei Paesi poco sviluppati e concorrono al mantenimento

L'aumento dei prezzi del cibo è stata infatti una delle cause che ha portato alle recenti rivolte avvenute nei Paesi del Nord-Africa e del Medio Oriente, rivolte che, quando hanno investito Paesi produttori di energie fossili, come nel caso della Libia, hanno prodotto reazioni a catena in quanto gli elevati prezzi delle derrate hanno spinto in alto i prezzi dei carburanti e questi, a loro volta, quelli degli alimenti, in un processo autosostenuto. L'industria agroalimentare, condizionata e condizionatrice dei nostri consumi, è sicuramente collegata con le problematiche di povertà e fame, ma non solo. La produzione agricola di tipo industriale, dominante nella nostra epoca, è generatrice di sempre più ampie deforestazioni, consumi idrici per la maggiore quota mondiale degli usi ed utilizzo di combustibili fossili in proporzioni impensabili (per muovere i macchinari, per produrre i diserbanti e fertilizzanti, per confezionare e trasportare in giro per il mondo il cibo). Tutto questo genera naturalmente esternalità esternalità negative per quanto riguarda l'effetto serra, l'esaurimento dei combustibili fossili, l'equità di accesso alle risorse alimentari nel mondo, il progressivo esaurimento di suoli fertili e delle risorse idriche, perdita di biodiversità anche di tipo alimentare, inquinamento diffuso e scarsa qualità degli alimenti, sia dal punto di vista del gusto che da quello della loro genuinità. Esistono molti modi per contrastare questo stato delle cose, primo fra tutti informarsi e crearsi una coscienza critica utile ad appoggiare con senso le nostre scelte individuali. Occorre scegliere, tra le tante vie del mangiare, quella più responsabile. Per esempio, aumentare il potere d'acquisto verso produzioni di tipo biologico, locale e di stagione; scegliere sempre frutta e verdura di stagione che, a differenza delle altre, consuma meno energia per essere trasportata e risulta più fresca e saporita;

Optare poi per alimenti biologici contribuisce a diminuire il consumo di combustibili fossili (utilizzati in larga misura per produrre diserbanti, pesticidi e fertilizzanti) e di emissioni in atmosfera di anidride carbonica, nonché a produrre alimenti più sani senza inquinare né impoverire la terra e le acque. Ridurre il consumo di carne, oltre ad apportare benefici alla salute, ostacola l'espansione dei grandi pascoli ottenuti dal disboscamento, favorisce una più alta produzione totale di cibo (una mucca per crescere necessita di tanta acqua e superficie di pascolo pari a quella utilizzabile per alimentare 8 persone con una dieta vegetariana) e limita le emissioni di metano in atmosfera prodotto dal sempre più alto numero di allevamenti presenti al mondo. mondo. Dinanzi alla necessità di introdurre nuove responsabilità sociali nelle relazioni economiche, determinante appare il contributo che l'agricoltura può dare, in quanto produttore di cibo, per la sua valenza territoriale e per le funzioni ambientali a cui assolve, oltre che per l'importanza che riveste come fonte primaria di reddito e cibo nei Paesi alle prese con le crisi economiche e politiche. Alla luce di queste brevi osservazioni, si richiede, quindi, che il Governo si attivi in Europa e nell'ambito delle relazioni internazionali per costruire una politica globale del cibo, che abbia finalità volte alla promozione dell'evoluzione culturale e politica, capace di dare nuovo valore e centralità al cibo come questione che riguarda non solo i produttori, ma l'insieme dei cittadini e delle comunità; che intervenga sui mercati finanziari orientandoli a proteggere un bene essenziale come il cibo dalle mire speculative; che guardi ai temi dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, della nutrizione e della cooperazione, superando le attuali divisioni; che favorisca il minore sfruttamento dell'ambiente nella produzione del cibo, insomma, che lavori per coltivare un mondo migliore. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud, alle mozioni presentate.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, le mozioni in esame intervengono su un tema molto delicato e importante che coinvolge e interessa il mondo intero. nel corso dell'illustrazione, è evidente che ancora oggi il problema della fame e della malnutrizione nel mondo non sia stato risolto e, soprattutto, come si sia ancora molto lontani dal raggiungimento di soluzioni idonee a sconfiggere questa piaga del nostro pianeta. L'agricoltura è sicuramente la fonte principale per la sopravvivenza delle popolazioni nei Paesi in via di sviluppo, ma è altrettanto vero che l'agricoltura intensiva, nonostante sia stata utile per sfamare la popolazione mondiale, è stata anche determinante per l'inquinamento di acqua, aria e suoli, per l'erosione della biodiversità e per la desertificazione delle terre. È ovvio che la constatazione di tale dato porti conseguentemente ad affermare che l'agricoltura intensiva non potrà più essere la strada da percorrere nel terzo millennio. Come osservato anche dalla FAO, per tutelare la popolazione futura sarà necessario, da un lato, aumentare la produttività, a causa della crescita esponenziale della stessa; dall'altro, utilizzare un modello produttivo più rispettoso degli ecosistemi nonché modificare le abitudini alimentari della popolazione, partendo da quelle dei bambini. I dati emersi dai numerosi studi sull'argomento sono allarmanti e indicativi di una situazione davvero molto complessa. Da un lato, infatti, è emerso che ancora oggi nel mondo soffrono la fame 925 milioni di persone e che il rischio maggiore per la salute degli individui è rappresentato dalla fame e dalla malnutrizione; dall'altro, circa per cento del cibo prodotto annualmente in tutto il mondo viene sprecato prima di essere consumato. Questo dato, nonché l'aumento dei prezzi delle materie prime agricole (determinato, come è emerso durante l'illustrazione delle mozioni, da numerosi fattori) sono indici eloquenti di come il problema della fame nel mondo non possa essere risolto soltanto attraverso il produrre di più. Il numero delle persone estremamente povere e prive di sufficienti mezzi di sostentamento rimane a livelli inaccettabili ed è sempre più evidente la diseguale distribuzione delle risorse alimentari tra Paesi ricchi e Paesi poveri. È assurdo, onorevoli colleghi, signora Presidente, vivere in un mondo che vede un essere umano su sette ridotto alla fame ogni giorno, pur vivendo in un mondo capace di nutrire tutti. Data la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite che, come noto, impegna, tra l'altro, gli Stati a sradicare la povertà estrema e la fame; riscontrati, sul fronte della lotta alla fame e alla povertà, i deludenti risultati del recente Vertice appurato che la situazione emersa tenderà ulteriormente ad aggravarsi, come indicato sia dall'OCSE sia dalla FAO, se non si determinerà una maggiore attenzione e senso di responsabilità della comunità internazionale, è ora che il Governo si impegni ad attivarsi sul fronte nazionale, in Europa e nell'ambito delle relazioni internazionali, al fine di far emergere la più ampia e condivisa determinazione per cercare di risolvere questa situazione, che,

Ho qui davanti a me una delle mappe della fame che si trovano su Internet - ce ne sono per tutti i gusti - da cui ho notato che il colore della fame attualmente è il *bordeaux*.

Certo, una qualche difficoltà a comprendere resta forte, se si accostano questi colori ad altre cifre che si sono lette in questi giorni.

Probabilmente, per chi come noi vive in una civiltà pervasa dal senso del diritto fino a poterla definire qualche volta saturata dallo succede che ci riesce forse difficile capire che la latitanza è maggiore dove se ne avverte di più il bisogno. Su questo, credo che si taccia abbastanza. Con Rodotà, penso si possa dire che non dovremmo mai stancarci di usare il linguaggio del diritto, e di usarlo come una opportunità di disciplinamento sociale.

Davvero le mozioni offrono tantissimi spunti. Sono stati quasi tutti sviluppati dai colleghi che mi hanno preceduto, e lo hanno fatto molto bene. bene. Per essere un po' meno edulcorati rispetto ad alcuni temi ancora presenti, converrà forse aggiungere che ci si dovrebbe impegnare comunemente per capire che molto c'è da fare ancora per superare una fase di tipo caritatevole, spesso affidata ad agenzie certamente nobili per finalità ma che non riescono a conseguire, secondo la mia opinione, quel risultato che dovrebbe essere conseguito in termini di maggiore coordinamento, di maggiore presenza, di una politica condivisa dei Paesi e degli Stati. Certamente, un ruolo del Governo non si può non declinare. Penso debba essere riconosciuta anche al nostro Paese la fatica di fare la sua parte. Siccome davvero il documento presenta tutte affermazioni condivisibili, pur nella loro semplicità, anch'io mi permetto di ricordare che tra le più semplici c'è anche una buona Dichiarazione fatta a Parigi nel

di far sì che tutti coloro che si impegnano in questi atti siano concordi, evitando duplicazioni, ridondanze e contraddizioni delle politiche supportate;

signor Sottosegretario, la mozione della Lega Nord (come le mozioni presentate dagli altri Gruppi parlamentari) tratta un argomento sicuramente complesso ed articolato, che da sempre vede coinvolti i Paesi industrializzati nel tentativo, sempre insufficiente, di aiutare i Paesi poveri (cosiddetto Terzo mondo). I numeri di chi, a tutt'oggi, non ha da mangiare a sufficienza sono impressionanti. Pensiamo al fatto che siamo nel 2011, che sono passati ben 42 anni da quando l'Apollo 11 sbarcò sulla luna, ma nonostante questi traguardi tecnologici

Sono numeri impressionanti, che tradotti in concreto ci portano a riscontrare che ogni cinque secondi nel mondo muore un bambino per problemi legati all'alimentazione. E questo non può che far riflettere tutti in maniera in maniera trasversale. Le zone geografiche maggiormente colpite da questo problema sono quelle in cui le condizioni climatiche non permettono di svolgere un'attività agricola redditizia. Parliamo quindi di alcune zone dell'Africa, per esempio il famoso Corno d'Africa, dove la siccità e la desertificazione non permettono, o permettono poco, di fare agricoltura. In alcuni Paesi (il Kenya, la Somalia e l'Etiopia,

chiaro che situazioni di questo genere non possono essere accettate al giorno d'oggi; bisogna quindi intervenire per migliorare le condizioni di vita di queste persone, che portano inevitabilmente, come conseguenze, a dei flussi migratori che sono spesso incontrollabili. Anche questi sono causa di tensioni internazionali, e in questi giorni ne vediamo gli effetti. Dobbiamo quindi intervenire in quei Paesi dove il problema è più rilevante: intervenire non solo economicamente, non solo finanziando questi Paesi, dove spesso i Governi e i governanti usano i soldi della cooperazione non si sa bene come, magari per acquistare armi con le quali assicurarsi il potere, ma operando per migliorare l'agricoltura, dando alle popolazioni locali una formazione culturale sulle nuove tecniche di coltivazione e fornendo loro la tecnologia adeguata al loro territorio di residenza. Ci sono realtà, oggi, che ci dimostrano che è possibile coltivare anche il deserto. Con il metodo dell'irrigazione goccia a goccia, gli israeliani, pur vivendo in una terra ostile dal punto di vista climatico (e non solo dal punto di vista climatico), riescono ad essere quasi autosufficienti dal punto di vista della produzione agricola, e a volte riescono anche ad esportare i loro prodotti agricoli. Serve quindi più razionalità negli interventi di cooperazione; serve, sì, finanziare gli interventi, ma questi devono essere di tipo politico e soprattutto tecnologico-politico. La diplomazia internazionale deve lavorare di più per portare più democrazia in questi Paesi, dove troppo territorio, troppe terre sono in mano ai latifondisti, che le usano e le sfruttano con monocolture, utilizzate poi dalle multinazionali per trarre il loro profitto. Ci deve essere maggiore frammentazione nella proprietà agricola per permettere a tutti di poter avere un pezzo di terra. Altro problema sono i troppi terreni utilizzati per produrre energia dall'agricoltura. Oggi è possibile puntare invece sulle energie rinnovabili e lasciare il terreno a disposizione degli agricoltori per produrre generi alimentari in grado di soddisfare le esigenze alimentari delle popolazioni residenti. Quindi, maggiore cooperazione, ma soprattutto più razionale e attenta utilizzazione delle risorse locali. È giusto aiutare queste persone a utilizzare correttamente i propri territori, migliorando le condizioni di produzione agricola, e quindi avere più cibo a disposizione; otterremmo condizioni di vita accettabili tali da permettere a quelle persone di rimanere nei loro territori di origine, evitando loro quegli inevitabili traumi conseguenti agli esodi forzati, cui assistiamo quasi quotidianamente in questi ultimi anni e a cui sono sottoposte le popolazioni in cerca di cibo e di lavoro. Aiutarli a casa loro non è un atteggiamento demagogico; pensiamo solo a quello che oggi è successo nel Nord-Africa, dove, a seguito dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari, in parecchi Paesi sono scoppiati disordini e guerre civili. È giusto aiutare queste persone, ma è giusto aiutarle a crescere culturalmente dando loro la possibilità di arrangiarsi e di essere autosufficienti. Se diamo loro qualche quintale di pesce risolviamo il problema dell'alimentazione per qualche giorno; se invece diamo loro una canna da pesca, una barca o una nave da pesca e insegniamo invece loro a pescare, risolviamo il problema per sempre. Questa non è demagogia, ma è il buon senso del nostro Gruppo della Lega Nord.

in un tempo nel quale si registra, piuttosto che una diminuzione, pure in passato preannunciata come obiettivo, un preoccupante ulteriore incremento del numero delle persone che nel mondo soffrono la mancanza di cibo (150 milioni negli ultimi due anni), il Gruppo del Partito Democratico ha avvertito la necessità di offrire il proprio contributo attraverso la mozione di cui sono primi firmatari i colleghi senatori Maria Teresa Bertuzzi e Roberto Di Giovan Paolo. Non è un caso che l'iniziativa sia partita da due sue espressioni che operano in ambiti e in Commissioni diverse e che, al di là della convinta sottoscrizione, quest'oggi siano intervenuti in discussione generale tanti colleghi del Gruppo del PD, la cui riconosciuta competenza sulle più disparate tematiche ha assicurato al dibattito una giovevole pluralità di apporti. In una materia tanto delicata e importante per i destini dell'umanità, è essenziale questo apporto multidisciplinare. Dico subito che sarebbe auspicabile anche da parte del Governo un'azione più interconnessa, chiamando in campo le diverse competenze di differenti Ministeri per mettere a punto una strategia vera e compiuta. A giudizio del Gruppo PD, è necessario insistere su due fronti per produrre più cibo laddove è più urgente: adottare politiche e programmi per assicurare sostentamento a milioni di poveri a rischio di inedia; promuovere misure per aiutare l'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo attraverso un potenziamento della produttività e un ampliamento della produzione, al fine di creare reddito e opportunità di impiego per le popolazioni rurali povere. In occasione delle ultime due Conferenze sulla sicurezza alimentare mondiale (giugno 2008 e novembre 2009), la FAO ha chiesto ai Paesi donatori di accentuare i propri interventi di assistenza e di valutare l'opportunità della riprogrammazione degli aiuti ai Paesi poveri penalizzati dal rialzo dei prezzi delle derrate. Il Partito Democratico, da subito, espresse condivisione della posizione della FAO, tesa, tra l'altro, a conseguire un effettivo rilancio dell'agricoltura quale principale strumento di lotta per combattere la fame nel mondo.

quell'anno, cioè quando il Governo Berlusconi era già in carica da alcune settimane. Oggi il Governo italiano è chiamato ad adoperarsi sia perché vengano onorati gli impegni sia affinché si individuino e si pongano in essere risposte più confacenti alle necessità vecchie e nuove.

È qui evidente l'esigenza di un cambio di marcia, a partire proprio da una diversa considerazione del ruolo che l'agricoltura può esercitare, non soltanto per la valorizzazione delle colture della terra e delle tipicità, ma anche quale leva di sviluppo nelle aree del Pianeta

o aggravino problemi alimentari per le regioni più povere. Vanno altresì tenute presenti le questioni relative alle variazioni demografiche, cioè all'incremento della popolazione mondiale, che da qui al 2050 toccherà picchi elevatissimi. Contestualmente a tale crescita, i cui indicatori già oggi si rilevano, siamo di fronte a decine e decine di milioni di nuovi poveri nel mondo. Anche e soprattutto per questa ragione, signora Presidente, vi è la necessità di un aggiornamento delle politiche al riguardo, affinché siano di lungo respiro e quindi capaci di intercettare le nuove emergenze e le straordinarie istanze che ne conseguono, oltre naturalmente agli interventi economico-finanziari ai quali di certo l'Italia non può sottrarsi. Infine, è urgente per noi sollecitare l'impegno della comunità internazionale affinché il tema della sicurezza alimentare divenga parte integrante delle politiche di sostegno che i Paesi sviluppati assumono a favore di quelli più poveri e svantaggiati, promuovendo così - per dirla con le stesse parole dei colleghi Bertuzzi e Di Giovan Paolo - una *governance* globale del cibo. È altrettanto urgente, però, che l'Italia compia uno sforzo di responsabilità ed assuma un ruolo di riferimento e di guida. A questi principi e agli obiettivi che ho tentato di sintetizzare si ispira la mozione alla quale il Gruppo del PD, mio tramite, annuncia il proprio voto favorevole. Esprimo altresì

che è la principale potenza ortofrutticola mondiale, ma riesce a trasformare o a conservare a malapena il 10 per cento della propria produzione ortofrutticola. significa che il 90 per cento della frutta e della verdura prodotte in India, che è un Paese immenso, quasi un continente, con più di un miliardo di persone, va disperso, distrutto. Potremmo continuare a lungo con altre affermazioni di questo tipo, ma non voglio ripetere le considerazioni, tutte interessantissime e dignitosissime, che sono state esposte oggi in quest'Aula dai miei colleghi.

tutti qui per sollecitare nuovamente il Governo a perseverare, continuare, accentuare il proprio impegno internazionale e multilaterale per affrontare e risolvere questo problema; non è vero

Semmai, è vero che l'Europa deve tornare ad essere protagonista del negoziato multilaterale per risolvere questi problemi. È vero che la FAO è importante, però è anche vero che, diciamo così, deve darsi una svegliata e diventare un organismo sempre più in grado di rispondere alle attribuzioni che le sono state affidate da parte dell'ONU e dei Paesi di tutto il mondo. la FAO - lo sappiamo tutti - è diventata un organismo che combatte la fame nel mondo portando a Roma molte persone del resto del mondo,

Ci deve essere quindi un impegno rinnovato, in questo senso, da parte del Governo, non tanto per riprendere i negoziati del WTO. Temo infatti che ormai il Doha Round sia fallito, perché ne sono venuti meno i presupposti.

dobbiamo liberarci da complessi di colpa nei confronti del mondo, che non dobbiamo avere, come quello sul protezionismo, che non applichiamo più. Dobbiamo invece essere consapevoli che possiamo fare molto di più come potenza agricola. Quindi, non carichiamoci di colpe che non abbiamo, di cui ci siamo liberati, e affrontiamo le sfide con coraggio e determinazione.

passare al punto successivo

Signora Presidente, mi sono iscritto a parlare per sollecitare

Signora Presidente, mi sono iscritto a parlare per sollecitare tutte le interrogazioni presentate al Ministero della giustizia dall'inizio della legislatura ad oggi, sia a mia prima firma che a prima firma della senatrice Poretti, tra le quali anche l'ultima, depositata ieri, relativa

sia che si trattasse di sovrappopolazione che dei numeri relativi agli agenti della Polizia penitenziaria, sia che si trattasse del trattamento riservato ai direttori

ha deciso di non fornire alcuna risposta a ciò che Marco Pannella denuncia da oltre 60 giorni (e da oltre 70 ore con uno sciopero prima dalla fame e adesso della fame e della sete) cioè l'illegalità patente delle istituzioni italiane nei confronti della nostra Costituzione e di tutti i trattati europei ed internazionali che l'Italia ha deciso di ratificare.

della nostra Repubblica (nel caso di specie, quello del Ministro della giustizia rispetto ai senatori della Repubblica) e, dall'altra, certifica ormai il totale distacco dal rispetto dello Stato di diritto. Concludo con un'altra citazione pannelliana: occorre stare molto attenti perché là dove vi è strage di diritto

penitenziari. Venerdì prossimo io sarò nel carcere di Torino, dove fortunatamente, solo perché vi sono grande partecipazione e presenza, cinque suicidi sono stati sventati nelle ultime settimane. Saranno sicuramente centinaia

Abbiamo già presentato un'interrogazione sulle gravi minacce rivolte, attraverso delle lettere, all'ex sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, il quale da tempo anima associazioni di volontariato su quel territorio che si battono ovviamente per la legalità. Ed è dell'altra notte la notizia di ulteriori intimidazioni, di attentati veri e propri effettuati su un bene confiscato alla camorra in un terreno nel territorio di Casal di Principe:

se continua così quel "modello Caserta" di cui il ministro Maroni e questo Governo tanto si sono vantati è destinato purtroppo al fallimento. Desidero ringrazio, inoltre, la magistratura e le forze dell'ordine per tutto

Signor Presidente, colleghi, poiché il Senato tra breve discuterà il proprio bilancio, sento il dovere - anche a nome del mio Gruppo di sollecitare il dibattito in Aula su di una questione di cui nelle settimane scorse ho già avuto occasione di attirare in via informale l'attenzione della Presidenza. Si tratta della questione dei dipendenti in soprannumero non effettivamente utilizzati dai Gruppi parlamentari. Con una delibera del Consiglio di Presidenza del 1993, aggiornata negli anni successivi con alcune altre delibere di contenuto analogo, è stato istituito un meccanismo volto a consentire ai dipendenti dei Gruppi parlamentari che risultavano non più costituiti

rispetto all'organico normale determinato in base al numero dei senatori. A tal fine la Presidenza del Senato allora dispose l'assegnazione a ciascun Gruppo a ciascun Gruppo di un contributo speciale, commisurato al numero dei dipendenti assorbiti. La stessa delibera disponeva altresì che il personale dei Gruppi disciolti che non fosse stato assorbito da alcun altro Gruppo, Gruppo, confluisse nel Gruppo Misto. Il risultato attuale del meccanismo descritto - di questo probabilmente la maggior parte dei colleghi senatori non è a conoscenza il Gruppo Misto si trova oggi ad avere formalmente alle proprie dipendenze un numero molto elevato di ex-dipendenti di altri Gruppi non più esistenti: un numero comunque fortemente sproporzionato rispetto alle dimensioni, alle esigenze operative e alle disponibilità logistiche dello stesso Gruppo Misto. Le sproporzioni, del resto, non riguardano soltanto questo Gruppo. A quanto mi risulta, la situazione è la seguente: il Gruppo del Popolo della Libertà dovrebbe, in base al numero dei propri senatori (131), secondo la regola generale, disporre di 21 dipendenti; ne ha invece 30; - il Gruppo del il Gruppo del Partito Democratico, composto da 106 senatori, dovrebbe disporre di 18 dipendenti; ne ha invece 24; - il Gruppo della Lega Nord, composto da 26 senatori, dovrebbe disporre di 9 dipendenti; ne ha invece 10; Gruppo dell'Unione di Centro, SVP e Autonomie, composto da 15 senatori, dovrebbe disporre di 7 dipendenti; ne ha invece 12; - il Gruppo dell'Italia dei Valori, composto da 12 senatori, dovrebbe disporre di 6 dipendenti; ne ha invece 12;

L'intera situazione merita una attenta riconsiderazione, non soltanto al fine di eliminare le sproporzioni evidenziate dai dati ora riportati, ma anche e soprattutto per verificare se e come il personale in soprannumero sia effettivamente utilizzato da ciascun Gruppo. Per quel che concerne, in particolare, il Gruppo Misto, risulta che ci siano diversi casi di persone che, pur ricevendo regolarmente da anni lo stipendio, tuttavia non mettono piede in ufficio. Più precisamente, risulta che siano a libro-paga di questo Gruppo i seguenti ex-dipendenti di Gruppi non più esistenti: 7 del Gruppo del Partito Socialista Italiano; 4 del Gruppo di Rifondazione Comunista; 3 del Gruppo dei Verdi; 2 del Gruppo della Democrazia Cristiana; 2 del Gruppo del Movimento Sociale Italiano; 1 del Gruppo del Partito Liberale Italiano;

13 delle 21 persone qui menzionate si trovano formalmente nella situazione di "dipendenti in soprannumero" del Gruppo Misto. Ma è certo che le persone "in soprannumero sostanziale" sono di più. Mi consta che tre di queste persone siano impegnate utilmente nella segreteria di altrettanti senatori. Delle altre, invece, non è dato sapere se, come e quanto esse siano oggi effettivamente utilizzate, e lo siano state nel corso dei diciotto anni trascorsi dalla prima delibera del 1993. La questione si pone anche perché non esiste presso il Gruppo Misto un posto fisico di lavoro ad esse riservato. Non mi è dato sapere se e quanto anche presso altri Gruppi si verifichino situazioni

con riferimento a quanto detto dal senatore Ichino, chiedo che questo argomento venga portato in Aula e con molta trasparenza si dia il giusto tempo per poter argomentare, e che quindi il testo consegnato venga conosciuto da tutti.

che hanno regolarmente assunto secondo le leggi del lavoro, i propri collaboratori, e si evince che ci sono anche senatori di serie A che utilizzano anche personale assunto a suo tempo dai Gruppi.

Penso ad esempio, al personale delle segreterie, spesso assunto e assegnato altrove, o al personale di cui alla delibera del 1993, non tutto presente presso i Gruppi, e senza una certa giustizia distributiva. Questo lo facciamo, cara Presidente e cari colleghi, nell'interesse della trasparenza del Senato, della dignità soprattutto del lavoratore e dignità della politica.

Avevo chiesto di parlare mentre il senatore Perduca, mi pare anche a nome della collega Poretti, svolgeva il proprio intervento. Al di là della sua formale richiesta di risposta alle interrogazioni, la mia sensazione è che in questa legislatura finora la questione delle carceri sia stata un po' monopolizzata esclusivamente nell'altro ramo del Parlamento, fin dall'annuncio di quel primo piano carceri, in occasione delle comunicazioni rese dal ministro Alfano, su cui poi si è improntata l'iniziativa della collega Bernardini alla Camera. Per tutta una serie di ragioni, anch'io, che ho presentato qui in Senato un disegno di legge su amnistia e indulto,

un approfondimento da parte del Senato di quelle implicazioni e di quei dati, sempre più drammatici, richiamati dal senatore Perduca, sui quali si sta svolgendo un dibattito pubblico, accentuato dallo sciopero della sete, da quattro giorni, di Marco Pannella, al quale non mi sento neanche in diritto di esprimere solidarietà; certo, ho profondo rispetto. A tal proposito, avrei preferito che quelle considerazioni avanzate ieri

Presidente, vorrei esprimere non soltanto in maniera quasi rituale e formale la solidarietà a Marco Pannella e al Partito Radicale tutto, ma anche l'apprezzamento, nei riguardi di Pannella e del suo partito, per l'impegno, la costanza e la serietà con cui stanno tentando da tempo di sottoporre all'attenzione generale un problema che è effettivamente esplosivo, quale il tema del sovraffollamento delle carceri, con tutte le implicazioni che esso prevede e comporta: e comporta: problemi di carattere sanitario, di promiscuità veramente incredibile, di invivibilità, di indecenza di condizioni, che sono disumane nel terzo millennio. È un problema grossissimo, ed è veramente sconcertante questo disinteresse generale da parte delle istituzioni, ma anche da parte dei mezzi di comunicazione, prima fra tutti la RAI. E bene avete fatto ieri a fare la manifestazione, che poca eco ha avuto rispetto all'intelligenza della manifestazione stessa. Vi siamo quindi grati per aver sottolineato la disattenzione del servizio pubblico - si fa per dire - radiotelevisivo rispetto ad un problema di così grave importanza. Io credo che tutti noi dobbiamo innanzitutto chiedere a Pannella di sospendere lo sciopero della sete: Pannella è indubbiamente una risorsa importantissima per tutti quanti noi. Ha sempre avuto il coraggio delle proprie azioni, fino in fondo, ed ha pagato anche con il suo coraggio e per il suo coraggio. Noi lo abbiamo apprezzato nel tempo quando facevamo parte di un partito, peraltro emarginato, e Pannella, attraverso anche Radio radicale, ci ha dato l'opportunità di avere una ribalta con la quale far conoscere le nostre idee e creare un dibattito politico. Di questo gli siamo grati: la nostra cultura di destra anche attraverso Radio radicale ha avuto la possibilità di avere una sua ribalta. Le chiediamo, Presidente, di intervenire fermamente per chiedere a Pannella di interrompere lo sciopero e chiedere anche autorevolmente, come lei sa fare, al Presidente del Senato di fare in modo che Pannella sia audito - faccio solamente un'ipotesi di intervento - in Commissione giustizia perché è giusto che esprima fino in fondo non solo le sue idee e le sue emozioni, ma anche le sue proposte. Ci affidiamo a lei e alla sua intelligenza politica, e crediamo di poter interpretare il sentimento comune di quanti semmai non condividono le idee di Pannella e dei radicali ma certamente ne apprezzano fin in fondo la importante azione politica.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche il mio intervento si colloca all'interno del drammatico tema della situazione penitenziaria. Intanto mi associo integralmente alle dichiarazioni della senatrice Poli Bortone relativamente all'invito rivolto a Marco Pannella affinché sospenda lo sciopero della fame, perché non è solo: non c'è bisogno di un ulteriore sacrificio che egli sta compiendo nelle sue condizioni fisiche perché, accanto a lui, all'interno del Parlamento, nella società civile ci sono tante persone che si battono per le sue stesse ragioni e per una maggiore dignità di vita all'interno delle carceri. Ciò detto, onorevole Presidente, purtroppo la drammaticità non cessa di attenuarsi. Walter Bonifacio ed Alessandro Giordano erano due detenuti del carcere di Padova, reclusi insieme ad un terzo carcerato. I primi due si sono suicidati: il primo il 24 maggio, il secondo nella notte tra il 5 ed il 6 giugno, entrambi utilizzando il gas. Questi episodi sono gli ultimi, purtroppo, di una lunga serie che nel decennio appena trascorso conta oltre 600 vittime. Ebbene, nonostante questo Parlamento più volte si sia occupato di temi legati alla detenzione, nonostante questo Parlamento più volte abbia approvato mozioni, ordini del giorno, atti di indirizzo e leggi, nonostante tutto questo, la situazione penitenziaria continua a non trovare uno sbocco, che non può essere circoscritto al dibattito di una giornata, ad un momento emotivo, alla denuncia di un episodio. È necessario un indirizzo forte affinché il tema entri nell'agenda del So anche che non è facile comprendere le ragioni dei reclusi, che vengono considerati quasi un non prodotto della nostra società, quasi degli alieni e invece non sono tali. Mi rendo conto che gli interventi che io e qualche collega facciamo spesso vengono considerati inopportuni e quant'altro, ma io intendo

colpevole l'atteggiamento del Governo della Regione, del Presidente della Regione, dell'assessore alla sanità e di quanti sostengono questa azione ignobile che sta facendo venir meno un diritto di tutti cittadini, soprattutto di quelli che sono privati della libertà.

Presidente, mi rivolgo a lei anche perché è persona sensibile. Pochi giorni fa ho ricevuto, oltre ad alcune *mail*, anche una telefonata di malati di SLA, o comunque malati con patologie con prognosi purtroppo infausta.

velocizzare la burocrazia, perché questi malati purtroppo hanno una vita molto breve. Uno di questi malati (io non riuscivo nemmeno a sentire per telefono cosa mi dicesse tanto era in condizioni precarie), nel richiedere l'invalidità e l'accompagnamento, ancora si è sentito dire nella commissione

presentiamo mozioni, cerchiamo di andare incontro a questi malati, però l'INPS con queste lungaggini darà l'accompagnamento e l'invalidità quando queste persone saranno decedute. La colpa è sempre e comunque della politica, però spesso - spero - in politica ci

ancora a queste persone vengono riconosciuti l'invalidità e l'accompagnamento dopo il decesso. Questa è una cosa veramente vergognosa! Credo che ci si debba attivare. Io presenterò un'interrogazione; quello che c'è da fare lo farò. Però, se c'è un presidente, ci sono dei nomi e cognomi, deve assolutamente farsi carico di queste procedure,

Signora Presidente, circa un mese fa, con i colleghi senatori della Sardegna, del Partito Democratico e della Commissione lavori pubblici, presentammo un'interrogazione circa il caso della privatizzazione della società Tirrenia di navigazione. A distanza di circa un mese (ed è normale in questo Parlamento, dove è difficile ascoltare la voce del Governo sugli atti di sindacato ispettivo), il Governo non ha detto niente, ma nel frattempo si sta combattendo sui mari nazionali del Mediterraneo, tra la Sardegna, la Sicilia, Napoli e Genova una vera e propria guerra; in ballo c'è il sistema dei trasporti marittimi del nostro Paese. Ad oggi le notizie sono che una vendita data per conclusa in una procedura di amministrazione straordinaria non è invece tale, perché i compratori contestano politiche di servizio pubblico della Regione autonoma della Sardegna ma non abbiamo nessuna parola ufficiale circa lo stato di questa vendita. Dietro la vendita non c'è solo la disponibilità di una flotta di navi e di servizi ai passeggeri alla vigilia della stagione estiva, ma anche un'accusa significativa all'*Antitrust* di

vorrei ricordarlo ai colleghi del Senato, non abbiamo un Ministro per le politiche comunitarie. Dopo le dimissioni del ministro Ronchi c'è il presidente Berlusconi, che sicuramente dopo ieri tornerà in Senato e ci racconterà quali sono le politiche del Governo nei confronti dell'Unione europea per garantire una situazione di sicurezza delle disposizioni disposizioni nazionali rispetto a questo tema.